L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea

Al fine di consentire un dibattito approfondito e di concludere le votazioni finali entro la fine della settimana medesima, il calendario prevede sedute, se necessario, fino a sabato mattina. La ripartizione dei tempi residui è stata rivista in seguito a cessioni concordate tra i Gruppi, fatte salve eventuali nuove armonizzazioni da parte della Presidenza. In coincidenza con il sesto anniversario della strage di Nassiriya, il calendario è integrato - giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 9 - con la discussione del disegno di legge per l'istituzione della Giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali per la pace, già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, il Governo e i Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno. Concluso 1'esame del provvedimento, riprenderanno le votazioni sul disegno di legge finanziaria. Il calendario della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 17 novembre, prevede al momento l'esame dei soli decreti-legge in scadenza, in materia di elezioni amministrative e di continuità del servizio scolastico. Nella mattina dì martedì 17 novembre sarà riconvocata la Conferenza dei Capigruppo per concordare eventuali ulteriori argomenti - compresi quelli fatti propri dai Gruppi di opposizione - da inserire nel calendario di tale settimana e di quella successiva.

per 1'adeguamento del Regolamento del Senato alla nuova normativa comunitaria derivante dalla prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge finanziaria. Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, avverto che con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno determinati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali. L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata preclusiva della discussione e della votazione di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati. Gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili. La valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame risulterà contabilmente nella Nota di variazione che il Governo presenterà al Senato subito dopo la sua approvazione.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.704 e 2.711, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti

2.194, 2.195, 2.457, 2.459, 2.473,

Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 2.704 e 2.711, sui quali il parere resta sospeso. La Commissione osserva, infine, che la proposta 2.716 risulta estranea per materia ai contenuti propri del disegno di legge finanziaria».

dall'operazione di cassa (chiamiamola così per non usare altri termini) che risponde al nome di scudo fiscale, di cui all'articolo 13-*bis*.

tutte le risorse derivanti da maggiori entrate sarebbero state utilizzate per l'attuazione della manovra di bilancio relativa agli anni 2010 e seguenti,

siano rivolte ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi a eventi celebrativi. Sempre nello stesso disegno di legge finanziaria, l'articolo 1, comma 4, prevede, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, la destinazione delle maggiori delle maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel corso del 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medi-bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti. È vero che noi siamo abituati ad una certa proliferazione di proclami e annunci, perché un giorno viene detto e scritto

ridotto il potere d'acquisto del reddito da lavoratore dipendente. Stiamo parlando di persone, di famiglie che vivono

dove, di fronte alla precarietà dei figli che, quando sono fortunati, hanno contratti a tempo determinato,

se la pressione fiscale fosse rimasta invariata dal 1980 ad oggi, ogni lavoratore avrebbe in busta paga 247 euro mensili in più.

una delle questioni fondamentali che il nostro Gruppo intende sottoporre all'attenzione dell'Aula. Dico subito che nel corso della discussione in Commissione e della discussione generale in questa sede

che pensano come noi che l'attuale patto di stabilità interno stia strangolando le capacità di investimento degli enti locali. Siamo in una fase particolarmente difficile della crisi economica e sociale che attraversa il nostro Paese.

Al momento attuale il patto di stabilità agisce impedendo a Comuni e Province di utilizzare le risorse che hanno a disposizione, per cui sono bloccati non solo gli investimenti futuri, ma anche i pagamenti degli stati di avanzamento delle opere già appaltate. Vi potete quindi immaginare quanto questo pesi negativamente sull'economia, tanto è vero che la questione è posta con forza non solo da noi noi e dai rappresentanti degli enti locali ma anche da tutte le rappresentanze economico-sociali del Paese. L'emendamento 1.0.5 si rivolge in modo particolare ai Comuni virtuosi, quei Comuni cioè che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2009 che presentano un andamento delle spese che mediamente sia inferiore a quello della media del comparto. L'emendamento L'emendamento tende a consentire a questi Comuni di fare i pagamenti in conto residui delle spese per investimenti;

i pagamenti, infine, per le spese di investimento nel campo dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. Si prevede anche un'altra fattispecie molto importante, che riguarda le opere assentite dal CIPE, che hanno già il finanziamento nazionale del CIPE, ma che per essere attivate necessitano di una quota di cofinanziamento locale. Siamo al paradosso che molti Comuni non possono spendere i soldi che hanno in cassa per questa quota di cofinanziamento, il che porta a bloccare anche importanti investimenti già decisi dal CIPE. Per questo, riteniamo molto importante che vi sia da parte della maggioranza e del Governo un segnale nella direzione delle questioni contenute in questo emendamento. che il Governo ha attivato un confronto con l'ANCI e che, non qui al Senato ma alla Camera, sarebbe disponibile ad apportare qualche modifica. mi appello alla maggioranza: credo che i senatori della maggioranza come noi non possano tornare sui loro territori senza avere una risposta positiva a questo punto: punto: dire di no qui al Senato a questa modifica significa pregiudicare anche il confronto in corso con l'ANCI e quindi possibili modifiche da parte della Camera. Per questo ci appelliamo alla maggioranza perché prema come noi sul Governo per ottenere su questo punto fondamentale una risposta positiva.

però a tutto c'è un limite. Nel momento in cui si pongono questioni di enorme rilievo, quali il patto di stabilità interno per gli enti locali e i molti altri argomenti affrontati da tali emendamenti, conoscere almeno il parere del Governo e della maggioranza, con poche parole ma in un modo comprensibile, credo sia non solo un diritto dell'opposizione ma un dovere di chi rappresenta il Governo e la maggioranza.

Ebbene, cari colleghi, se esso non venisse approvato ho l'impressione che invece di chiamarlo patto di stabilità dovremmo chiamarlo patto di assurdità.

sulle spese in conto capitale: si tratta quindi di impegni già assunti e di soldi che già ci sono nelle casse di Province e Comuni. Da una parte, diciamo che la pubblica amministrazione non paga le imprese, poi, però, imponiamo con il patto di stabilità che, per rispettare la norma, gli enti locali siano costretti a non pagare le fatture che arrivano relativamente agli investimenti. La seconda questione che viene posta è la possibilità di sbloccare i fondi per gli investimenti per mettere a norma le scuole, per mettere a norma il dissesto idrogeologico del nostro Paese. Ci lamentiamo quando ci sono

In quest'Aula, quindi, ci sono forze potenzialmente maggioritarie che chiedono al Governo di cambiare l'assurdità di questo patto che strangola gli enti locali e l'economia italiana.

- proporre un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare i termini del patto di stabilità interno entro la fine dell'esame parlamentare della finanziaria. È infatti veramente assurdo procedere in questo modo e impedire ai Comuni italiani di avere ciò che è dovuto e richiesto da tutte le imprese, ovvero semplicemente la possibilità di spendere i soldi che hanno in cassa per fare investimenti. In quest'Aula ci sono forze anche della maggioranza che sono d'accordo con noi; chiedo quindi che si esprimano affinché sia possibile arrivare almeno ad un ordine del giorno che abbia queste caratteristiche.

Dichiaro aperta la votazione.

nel senso che ai Comuni virtuosi non è permesso utilizzare gli avanzi di bilancio per i propri lavori e per i lavori socialmente utili. Io non capisco come alcuni membri della maggioranza, ad esempio gli amici della Lega Nord, possano votare contro un emendamento di questo tipo. Al relatore faccio presente che l'anno scorso lo stesso emendamento aveva avuto, se non altro, il diritto ad essere trasformato in una raccomandazione. Ciò non è servito a nulla ma, almeno, l'anno scorso il parere non era stato negativo. Chiedo la votazione

sono concentrati su alcune tematiche che noi riteniamo essenziali ed hanno contenuto diverso. Uno degli emendamenti più importanti - il 2.7 - riguarda l'utilizzo in forma strategica strutturale per la nostra economia del credito d'imposta, in modo particolare utilizzandolo come strumento compensativo per le condizioni di svantaggio delle imprese nel Mezzogiorno, essendosi registrato, rispetto a una iniziativa in sede legislativa assunta dalla Regione siciliana, il via libera dell'Unione europea, alla quale il provvedimento è stato notificato. L'Unione europea ha considerato valido questo strumento di incentivazione allo sviluppo;

per quanto concerne l'incentivazione allo sviluppo nel Mezzogiorno. Tale strumento è stato poi sostanzialmente abbandonano a causa di una riduzione drastica del finanziamento della mancanza di qualsiasi alternativa dal punto di vista dello stimolo all'impresa, con misure differenziate sul territorio nazionale. Rispetto al grande tema dello sviluppo del Mezzogiorno, riteniamo che il Governo, che ha preannunciato un piano straordinario, debba superare la fase degli annunci e presentare un pacchetto di misure concrete, a cominciare di quelli che immaginiamo siano strumenti verificati e positivi, come il credito d'imposta, strumento che consideriamo tra l'altro quale anticipazione di un meccanismo più radicale,

stimolo, non soltanto per l'impresa autoctona del Mezzogiorno, ma anche per una delocalizzazione, all'interno del territorio nazionale, di tante aziende del Nord del Paese, al fine di garantire al sistema Italia il recupero di un'area straordinariamente importante, qual è il nostro Sud, nell'interesse dell'economia nazionale. Rispetto alle tante analisi e ai tanti commenti dei mesi scorsi su come dovrebbe essere realizzato questo intervento straordinario nel Mezzogiorno,

presenza dello Stato incisiva ed impegnativa in relazione ad una delle precondizioni assolute per lo sviluppo, che è la legalità sul territorio. vorremmo che il piano di infrastrutturazione straordinaria, che è parte del programma di Governo, venisse varato compensando l'abbandono di politiche di intervento sulle infrastrutture, che si

ed un meccanismo di automatismo che dovrebbe eliminare qualsiasi intermediazione. L'adozione di questo meccanismo di carattere generale nel Mezzogiorno assumerebbe un valore in più rispetto al tema della legalità e alla funzione spesso frenante e corruttiva della pubblica amministrazione.

all'intero territorio nazionale, sia specificamente alla Regione siciliana. In questo senso, immaginiamo di poter utilizzare la forza finanziaria irrigidita della Cassa depositi e prestiti,

particolare emergenza in queste settimane, ma anche un piano strategico per l'intero Paese, utilizzando la Cassa depositi e prestiti. Ancora, vorrei tornare sulla annosa questione delle accise sui prodotti raffinati in Sicilia. Nel nostro Paese, vi sono aree geografiche che per ragioni legittime, essendo di confine, godono di trattamenti speciali relativi alla materia

imprese, conosce soltanto danni gravissimi: inquinamento e anche gravi patologie che sono state verificate in termini epidemiologici da ricerche scientifiche di assoluta serietà. Da tempo, almeno dal quest'Aula proponiamo diverse misure che consentano di ristorare in modo dignitoso quei territori che sopportano, nell'interesse dell'intero Paese, questo tipo di impianti.

Questa norma ha conosciuto il consenso bipartisan a fasi alternate: quando la proponemmo nel 2006, la votava il centrodestra contro il Governo di centrosinistra, quando l'abbiamo proposta nel 2008 l'ha votata il centrosinistra contro il Governo di centrodestra. Se per una volta la votassimo secondo convinzione, per il buonsenso che essa porta essa porta in sé e per la giustezza delle ragioni che la assistono, avremmo compiuto un atto politicamente anche logico e coerente. Per quanto riguarda il Movimento per le Autonomie, questa vicenda delle accise rimane una partita aperta che abbiamo, tra l'altro, chiesto al Governo di affrontare in sede di legge delega sul federalismo fiscale e dove un via libera in linea di principio è giunto.

in questa finanziaria dia un segno di attenzione serio al Movimento per le Autonomie e al suo contributo leale alla maggioranza; la nostra è una lealtà che non può essere acritica, e ovviamente la disattenzione verrebbe considerata un fatto politicamente non irrilevante.

ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (TIA), essendo una tassa e non una mera tariffa, non è soggetta ad IVA, e quindi non è dovuto quel 10 per cento applicato fino ad oggi e impropriamente pagato dai contribuenti. Non è una cifra simbolica, se si pensa che una famiglia paga in media 120 euro l'anno per il ritiro e lo smaltimento della spazzatura e che in Italia ci sono 18 milioni di famiglie che praticamente hanno pagato una tassa sulla tassa. Non solo: 1.200 sono i Comuni interessati e le aziende di gestioni che ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica, che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro. Il PD ha quindi previsto alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che mirano ad evitare, da una parte, il caos burocratico-amministrativo e, dall'altra, che il peso dell'indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio o, peggio, che non venga realizzato il diritto del cittadino ad essere risarcito. Chiediamo quindi, attraverso l'emendamento 2.95, di risarcire il cittadino dell'indebito, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a circa 150 milioni di euro. Chiediamo anche, con l'emendamento 2.287, che gli eventuali maggiori oneri a carico dei Comuni che sono assimilabili a sostituto d'imposta siano a carico della fiscalità generale fino a quando non si disciplinerà in maniera puntuale puntuale la normativa al riguardo. Attraverso l'ordine del giorno chiediamo che il Governo su questo tema emani in tempi brevi brevi apposite disposizioni normative interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando così di lasciare le aziende di erogazione del servizio e i Comuni

è però rimborsare al cittadino il pagamento di una tassa che è stata pagata, di una tassa su una tassa. È corretto quindi che il cittadino venga rimborsato almeno di questo, in attesa di chiarimenti dal punto di vista legislativo*.

L'emendamento 2.53 reintroduce le agevolazioni contributive che erano state previste dalla legge n. 67 del 1988, determinandone un incremento. Questo riguarda sia i territori montani, per i quali è previsto un adeguamento della aliquota al 75

oggettivamente rispondono ai requisiti di aree svantaggiate, come Abruzzo, Molise e Basilicata.

per quanto riguarda il sostegno al reddito delle migliaia e migliaia di imprese agricole: l'aumento dei costi e il crollo dei prezzi all'origine stanno mettendo in ginocchio centinaia di migliaia di famiglie di agricoltori. A questo la politica del Governo non è stata di grande aiuto. La finanziaria 2009, lo ricordo a me stesso, ha eliminato le agevolazioni contributive per la manodopera agricola.

anche perché non ci convince la proposta avanzata dal ministro dell'agricoltura Zaia circa il fondo di ripartizione previsto dall'articolo 68 del Regolamento CE, nel quale lui orienta i maggiori investimenti sulla filiera del tabacco e sulla zootecnia, cioè su settori dell'agricoltura

di persone portatrici di handicap. Nel caso in cui il relatore ed il Governo ritenessero di non poter accogliere l'emendamento, proporrei la sua trasformazione in un ordine del giorno. Ne approfitto per illustrare anche l'emendamento 2.115, che prevede un'incentivazione fiscale per l'acquisto di biciclette. Il Governo ha recentemente assunto un'iniziativa molto positiva,

2.149 provvede a prorogare fino a tutto il 2010 la detrazione IRPEF del 19 delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L'agevolazione, in base alla legislazione vigente, è prevista fino a tutto il 2009, per una spesa massima di 250 euro a persona. L'emendamento 2.151 mira a colmare un'ingiustizia conseguente ad un vuoto legislativo. La legge n. 448 del 2001 prevedeva la possibilità per l'acquirente di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato, oggetto di restauro o ristrutturazione edilizia, di detrarre dall'IRPEF parte del valore degli interventi eseguiti. Queste detrazioni sono state negli anni prorogate, tranne però che per gli interventi di ristrutturazione avvenuti nel 2007. che se la compravendita riguarda un immobile facente parte di un edificio ristrutturato nel 2007, e solo in quell'anno, l'acquirente non ha diritto di beneficiare della detrazione. chiede la proroga per il triennio 2010-2012 della disposizione, introdotta dalla finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 335, per quanto riguarda i costi riferiti all'immobile strumentale del professionista. In tal modo si dovrebbe concedere la possibilità agli studi professionali di dedurre le quote di ammortamento o dei canoni di locazione, finanziare gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione acquistati dai professionisti stessi fino al 31 dicembre 2012. Si tratta di un intervento volto ad assimilare la disciplina fiscale del professionista a quella delle imprese. L'emendamento 2.177 provvede a prorogare anche per il 2010 a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, la detrazione IRPEF del 19 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione, ed effettivamente rimaste a proprio carico. L'emendamento 2.178 provvede a prorogare a tutto il 2010 la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Questo è un emendamento importante - lo dico anche ai senatori della maggioranza che scade a fine 2009 la norma che agevola gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, legandoli al bonus sulle ristrutturazioni immobiliari. La norma che si intende prorogare, così com'è stato fatto nella presente finanziaria per le ristrutturazioni immobiliari,

poiché riguarda gli interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociale e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche anche per combattere l'inquinamento. Infine, l'emendamento 2.554 è volto a rendere stabile il meccanismo del 5 per mille a decorrere dal 2010. Ricordiamo che il 5 per mille serve a finanziare le organizzazioni *no profit* che operano nel sociale. Le risorse fino ad oggi stanziate valgono solo fino al 2009; il 2008 deve ancora essere pagato,

Il Ministro ha indicato questa posta tra quelle meritevoli di essere rifinanziate nella cosiddetta fase 2 della manovra, ovviamente se si troveranno le risorse necessarie.

il problema della conciliazione e della condivisione. Si tratta di questioni che abbiamo posto in numerose altre occasioni come sollecitazione al Governo. Ci saremmo aspettati che, nei numerosi decreti che il Governo ha presentato in Parlamento, fosse inserita qualche misura a favore dell'espansione del lavoro femminile e della conciliazione, ma niente è successo. Ci siamo scontrati con una sordità assoluta; abbiamo registrato soltanto annunci per un futuro indeterminato e indefinito. I nostri emendamenti partono dalla cruda realtà, ossia dalla crisi economica che stiamo vivendo: è infatti noto che la crisi colpisce soprattutto le donne e lo fa in varie forme. Partono anche da alcune analisi che gli osservatori unanimemente ci consegnano, innanzitutto dal fatto che il lavoro femminile costituisce uno straordinario valore per lo sviluppo, un valore civile che attiene alle eguali opportunità fra uomini e donne.

Siamo molto al di sotto della media europea, ossia a un insopportabile 31 per cento nel Mezzogiorno. Il lavoro femminile ha anche un valore sociale, perché si sa che a un maggiore tasso di occupazione femminile corrisponde una maggiore coesione sociale, una maggiore serenità delle coppie e delle famiglie e, di conseguenza, una crescita della natalità, che è ancora a un tasso poco sopra lo zero nel nostro Paese, anche a causa dell'incertezza sul futuro. Soprattutto, il lavoro femminile rappresenta un valore economico. Voglio riportare un dato: ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro, si creano 15 nuovi posti di lavoro. Se lavorassero tante donne quanti sono gli uomini, il nostro prodotto interno lordo crescerebbe del 17,5 per cento. Pertanto, il lavoro femminile è uno straordinario fattore di sviluppo per l'intero Paese.

La seconda concerne l'imprenditoria femminile, prevedendo sostegni e facilitazioni soprattutto all'accesso al credito, perché questo è il maggiore problema che le imprenditrici incontrano nella loro attività.

Il tema che affronto è quello del cumulo delle contribuzioni nelle opere di ristrutturazione edilizia. Io credo che anche gli episodi tragici di queste ultime settimane e giorni (penso, ad esempio, ai tragici fatti di Ischia) impongano una riflessione sull'opportunità

Nondimeno, ritengo assolutamente complementare a quanto ho detto anche l'intervento dei privati, che debbono avere la possibilità di godere di incentivi per poter riqualificare i propri immobili. finanziaria prevede la proroga delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, ma non stabilisce ancora il cumulo di queste agevolazioni con quelle indirizzate all'efficienza energetica, alla sicurezza e al recupero delle tipologie tradizionali, così importanti soprattutto nel grande patrimonio storico delle nostre città. L'ordine del giorno vuole pertanto invitare il Governo a prendere in considerazione l'opportunità di attivare un meccanismo di cumuli

privata, che è stato oggetto di riflessione in altre circostanze e che ha impegnato quest'Aula e il Governo a cercare di reperire le risorse necessarie per sostenere un settore, che vive un momento particolare per la sua trasformazione dal punto di vista tecnologico e anche in ordine alla necessità di compiere investimenti per costruire un pluralismo informativo nel nostro Paese. Per queste ragioni, insisterò affinché il Governo si faccia carico di questa tematica.

dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012: si tratta, complessivamente, di 3.594 milioni per il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui 1.278 per i per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Le cifre stanziate dal Governo all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria sono davvero irrisorie, di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale. sulla base di quanto stabilito nel comma 16, non vi è poi alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e di conseguenza del rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego. In base al comma citato, infatti, tutto ciò viene rinviato alla successiva definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione.

ai lavoratori del pubblico impiego la fruizione di un'indennità maggiore, pur tenendo conto della ricerca di un equilibrio nella finanza pubblica. L'emendamento 2.274 contiene un altro intervento per rendere compatibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

quindi che il Governo adotti ogni intervento utile al rilancio delle politiche a sostegno dell'occupazione e al reddito e quindi chiediamo di aumentare le somme a disposizione per il Fondo per l'occupazione. l'emendamento 2.272 chiediamo il riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione e quindi l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria. Speriamo che questi emendamenti possano essere accolti anche dalla maggioranza, vista la grave crisi economica in cui versano tante famiglie italiane. *(PD)*. Signora Presidente, intendo illustrare in particolare l'emendamento 2.253. Il ministro Maroni ha negato per mesi e mesi l'esistenza di tagli alla sicurezza. Ha ammesso tale situazione solo all'indomani della manifestazione unitaria di tutti i sindacati della polizia, sostenuti ed appoggiati dai COCER delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Ancora, nei giorni successivi il Ministro dell'interno si è detto pronto a votare, se presentate, eventuali proposte dell'opposizione per garantire più sicurezza. Ecco, signora Presidente, le proposte ci sono e sono contenute. Per quello che riguarda le risorse contrattuali da destinare al comparto della sicurezza e della difesa, in questo emendamento si prevede infatti di raddoppiare lo stanziamento per il rinnovo del contratto di questi lavoratori che, oltre a svolgere una funzione fondamentale nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, rappresentano inequivocabilmente un settore di eccellenza della pubblica amministrazione. Attendiamo quindi che il Ministro dell'interno sia coerente e conseguente con le proprie dichiarazioni, svolgendo la necessaria azione persuasiva sia nei confronti dell'intero Governo che del suo Gruppo di riferimento. Il Ministro e la maggioranza non si illudano di risolvere questo problema con le parole o le promesse. Infatti, da tutti deve essere attentamente valutato il giustificato malessere presente tra il personale delle forze di polizia e delle Forze armate per le condizioni in cui è costretto ad operare, anche a causa dei tagli lineari apportati ai fondi per l'esercizio e alle risorse per il reclutamento. Allo stesso tempo si tratta di considerare la situazione che si è andata consolidando in questi mesi, ovvero che cosa significhi per gli operatori della sicurezza anticipare di tasca propria le spese di viaggio quando si è comandati in servizio fuori sede, o quando non ci sono i soldi per pagare l'affitto del commissariato dove si presta servizio, o quando le volanti non possono uscire perché non c'è benzina e per lo stesso motivo rimangono in porto le navi della Marina militare, restano a terra gli aerei dell'Aeronautica, vengono annullate le esercitazioni addestrative delle forze di terra. In ogni caso, rammento all'Aula che nella manifestazione del 28 ottobre non era secondaria la questione dei rinnovi contrattuali. Stiamo parlando di circa 500.000 persone, l'80 per cento delle quali percepisce redditi medio-bassi. Sono lavoratori, donne e uomini, ai quali affidiamo il rispetto della legalità, la sicurezza dello Stato e la difesa della pace in Italia all'estero. A chi antepone, signora Presidente, a questa discutibile situazione l'esigenza di una razionalizzazione del settore, rispetto alla quale siamo prontissimi a confrontarci in Parlamento, diciamo con altrettanta chiarezza che non si può far pagare al personale il prezzo di riforme da fare e che vengono continuamente rinviate. *(Applausi

e 2.575. Quanto al Piano straordinario di edilizia pubblica, l'articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra di esse spicca il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratifica ai sensi della legge 25 ottobre 1977, In particolare, è norma di legge dello Stato italiano l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che prevede che gli Stati riconoscano il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguato, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Troppo spesso il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha palesato preoccupazione nei confronti del *modus operandi* dello Stato italiano, che sembra non accettare ancora che alcuni diritti economici, sociali e culturali, vengano accolti. Il Comitato ha espresso perplessità anche per il continuo aumento degli affitti, la privatizzazione dell'edilizia popolare ed il *deficit* di edilizia sociale per le famiglie a reddito basso. La spesa statale in materia di edilizia residenziale è prevalentemente indiretta, cioè delegata a soggetti pubblici quali gli enti locali, ma il processo di decisione, dalla pianificazione all'attuazione, è statale e non appare strutturato per dare un contenuto di efficienza ed efficacia a tale delega. Le decisioni di investimento sono abitualmente assunte sulla base di accordi tra amministrazioni senza il supporto della valutazione economica che, invece, dovrebbe essere introdotta già nella fase di pianificazione, seguendo linee guida obbligatorie, standardizzate e metodologicamente solide, in modo che il soggetto finanziatore - il Ministero delle infrastrutture - possa confrontare progetti concorrenti, definire le conseguenti priorità in modo trasparente ed adottare scelte razionali. Complessivamente prevale, a nostro avviso, una logica di processo piuttosto che di risultato: gli obiettivi dei diversi programmi di spesa ed i risultati attesi non sono chiaramente individuati e gli indicatori per misurarli non sono adeguatamente definiti e quantificati. Preliminare, tuttavia, ad un diverso processo pianificatorio in materia di edilizia residenziale è lo stanziamento di risorse necessarie per far fronte alle esigenze abitative della popolazione meno abbiente. In questa già critica situazione il Governo ha, invece, scelto di apportare una variazione negativa agli stanziamenti previsti per il Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica. Con l'emendamento 2.340, al fine di compensare la suddetta variazione negativa, l'Italia dei Valori auspica l'incremento di 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. L'emendamento 2.377 fa invece riferimento al Fondo per gli interventi straordinari. Alla luce di recenti stime, in Italia ci sarebbero non meno di 80.000 edifici pubblici da consolidare e mettere in sicurezza. In particolare, circa 22.000 edifici scolastici sono in zone sismiche, 16.000 in zone ad alto rischio e circa 9.000 non sono costruiti con criteri antisismici moderni. criteri antisismici moderni. Dall'evento sismico che ha così tragicamente colpito l'Abruzzo è emerso un imperativo categorico: provvedere alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici, officine del sapere dei nostri giovani, come ha tante volte ribadito il senatore Astore nei suoi interventi. È inaccettabile che lo Stato, quasi fosse un Giano bifronte, imponga ai propri imprenditori di garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro (il pensiero corre al decreto legislativo n. 81 del 2008) e poi sia il primo a sottrarsi davvero a tale dovere. È inaccettabile che dopo i ripetuti e drammatici casi di crollo di edifici scolastici vi siano ancora scuole che non siano messe in sicurezza statica per mancanza di stanziamenti. proporre di incrementare di 25 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con decreto-legge 30 settembre 2003, Il suddetto Fondo è volto a contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte. Alla luce dei drammatici fatti verificatosi che hanno palesato l'inadeguatezza delle nostre infrastrutture a fronteggiare il rischio sismico, si auspica il suddetto incremento al fine di realizzare interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione e mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti ove sottoposti a rischio sismico o idrogeologico.

In particolare, si incrementa di 7 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 lo stanziamento previsto nell'ambito della missione diritto alla mobilità, programma sviluppo e sicurezza del trasporto aereo»

Il Piano generale della mobilità, riportato in sintesi nel DPEF 2008-2011, nel capitolo «Mobilità» prefigura azioni per realizzare un sistema di trasporti sicuro, efficace e sostenibile, enunciando i seguenti obiettivi su cui riprogrammare le scelte degli interventi sulle reti infrastrutturali: Mediterraneo e autostrade del mare; intermodalità, sia sotto il profilo del sostegno alle imprese per il combinato ferroviario e marittimo, sia con la realizzazione di interporti; politiche di sostegno alla portualità, attraverso servizi intermodali e piattaforme logistiche retroportuali, realizzazione di grandi porti di *trans-shipment*; trasporti sostenibili, con l'affidabilità dei servizi e dei diritti dei passeggeri; incremento dell'efficienza energetica e della propulsione ecocompatibile; riduzione dell'inquinamento ambientale; servizi di qualità per i passeggeri. All'uopo, si auspica l'incremento di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 del Fondo perequativo a favore delle autorità portuali. Concludo illustrando l'emendamento 2.575, che attiene allo sviluppo del trasporto pubblico locale, argomento che riteniamo molto importante. L'assetto dei servizi pubblici locali, in particolare del trasporto, è da sempre oggetto del dibattito economico e politico. Il servizio di trasporto pubblico locale incide trasversalmente sulla vita dei cittadini, in particolare sul potere d'acquisto delle famiglie, sulla qualità dell'ambiente e sulla competitività delle imprese italiane.

L'articolo 16 della Costituzione sancendo che «Ogni cittadino può circolare (...) liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (...)», configura un diritto alla mobilità, ponendo in capo allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto che lo rendano effettivo.

all'inadeguatezza del sistema infrastrutturale. Appare necessario adottare una politica programmatica di lungo periodo, al fine di incrementare la fruizione del trasporto pubblico locale, di migliorare la vivibilità dei tessuti urbani e la qualità dell'ambiente. Occorre, inoltre, conferire centralità alle specificità territoriali ed agli elementi di sostenibilità finanziaria ed ambientale dei progetti. Nonostante le condizioni in cui versa il nostro sistema di trasporto pubblico locale, il Governo ha deciso di ridurre e tagliare i finanziamenti.

il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. In particolare, si incide nell'ambito della missione diritto alla mobilità, programma sviluppo della mobilità locale.

nei giorni scorsi il sottosegretario Giovanardi ha lamentato il fatto che in questa finanziaria avremmo avuto meno attenzione dell'anno scorso alle politiche per la famiglia. Sempre nelle settimane scorse anche il ministro Sacconi e altri esponenti del Governo hanno ammesso che il *bonus* per le famiglie e la *social card* non sono riusciti a raggiungere i destinatari: solo il 40 di essi sono stati raggiunti e soprattutto non si è riusciti a raggiungere quei destinatari, come le famiglie con figli, che sono maggiormente toccati dalla crisi. In effetti, nel Sud le famiglie con figli sono impoverite ulteriormente e abbiamo il tasso di povertà minorile più alto d'Europa. durante questa discussione sarebbe stato opportuno fare un bilancio delle politiche del Governo sulla *social card* e il *bonus* per le famiglie, come è stato ammesso dai Ministri, e forse cercare di rettificare questa politica perché, se non abbiamo più dei fondi, abbiamo dei fondi che non sono stati spesi perché i destinatari non sono stati raggiunti o lo sono stati malamente, i problemi si aggravano. Quindi decidiamo oggi se vogliamo ripristinare un

Partiamo dal presupposto che, per esempio, in Europa si spende una media di 2,5 del PIL per l'autosufficienza e in Italia solo lo 0,12. Un secondo emendamento riguarda l'aumento degli assegni familiari, che dovrebbero cercare di aiutare le famiglie maggiormente impoverite in termini assoluti e di impoverimento delle opportunità.

le case famiglia. Ho visitato, come molti di voi, molte case alloggio; soltanto a Palermo ne ho visitate una decina e due di queste hanno chiuso perché il Comune di Palermo non sostiene le case famiglia.

intervengano a sostenere le case famiglia dove vivono bambini abbandonati o bambini che versano in condizioni molto delicate (perché abbandonati

pertanto alla Commissione e al Governo che, almeno su alcune questioni, si possa intervenire positivamente. l'emendamento 2.332a si riferisce ad un'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per sostenere le scuole non statali che svolgono una funzione educativa riconosciuta nel nostro Paese. L'emergenza educativa richiamata ancora ieri dai vescovi italiani rappresenta un problema centrale della famiglia e delle nostre famiglie.

la Presidenza continua a ricevere richieste di intervento da parte di colleghi che sono già stati invitati ad illustrare i propri emendamenti e ordini del giorno. In spirito di collaborazione, la Presidenza darà la parola ai senatori che l'hanno richiesta ma invita, al tempo stesso, a una maggiore attenzione per garantire un ordinato svolgimento dei lavori.

Presidente, volevo illustrare l'emendamento 2.367 che attiene ad un provvedimento sul quale alcune finanziarie si sono già soffermate e sul quale chiediamo anche al Governo di porre attenzione. In particolare, si tratta delle vittime del dovere e della criminalità. Sappiamo che su questo punto molte disposizioni si sono ripetute negli anni. In questa finanziaria, attraverso questo emendamento, chiediamo che si sanino questioni pregresse per quanto riguarda le vittime del dovere e della criminalità, atto doveroso che spesso questo Governo ha detto di voler compiere. Per questo invito tutti i colleghi a porre attenzione a questo emendamento, perché credo che sarebbe un gesto doveroso da parte del Senato.

Signora Presidente, non intervengo sugli emendamenti da me presentati in materia di giustizia, che peraltro si illustrano da soli, stante i tagli costanti che sono stati operati; vorrei invece illustrare tre emendamenti ed un ordine del giorno in materia di amianto. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.11, 2.457, 2.411 e dell'ordine del giorno G2.124.

per meglio dire un'interpretazione autentica, rispetto al Fondo per le vittime dell'amianto istituito con l'ultima finanziaria del Governo Prodi.

degli uffici aperti al pubblico che sono inquinati da amianto. Ricordo, e concludo, che si tratterebbe di un atto di giustizia e per questo proponiamo la trasformazione anche di questo

di un emendamento importante, che consente il recupero di circa 40 milioni di euro già stanziati a favore dell'assunzione di nuovi ricercatori. Alla fine Alla fine del 2006, con la legge finanziaria 2007, sono state stanziate all'articolo 1, le seguenti cifre per l'assunzione di ricercatori: per l'anno 2007, 20 milioni di euro; per l'anno 2008, 40 milioni di euro; per l'anno 2009

nostra struttura di ricerca, stanno guardando con attenzione. tediarvi con la tecnicalità abbastanza complessa con cui viene recuperata la possibilità di utilizzare le risorse stanziate per il 2009 a partire dal 2010 per questi ricercatori; ma si tratta di un emendamento che favorisce la nostra ricerca, ha un'entità importante (40 milioni di euro circa) e

Come viene puntualmente indicato nell'ordine del giorno, vi è la necessità di destinare risorse adeguate, quantomeno corrispondenti a quelle già esistenti, al sostegno degli interventi previsti dalla legge n. 431 del 1998. Ciò non riguarda più solamente le famiglie delle fasce più deboli, ma gli effetti della crisi economica hanno iniziato ad avere pesanti ripercussioni anche sulle famiglie del ceto medio, che non riescono a far fronte alle spese per l'affitto o non riescono più a trovare un altro alloggio nel caso in cui debbano lasciare quello nel quale abitano. L'emergenza abitativa, lungi dall'essere risolta, sta invece rivelandosi ancora più estesa e drammatica di quanto si possa percepire; i sindaci sono in prima linea ad affrontare un problema sociale per il quale non possono essere ridotte le risorse, proprio in questa fase di crisi occupazionale e di riduzione dei redditi disponibili di molte famiglie, soprattutto con figli, con persone anziane e con persone disabili a carico. Il Governo ha il dovere di prevedere un sostegno adeguato e concreto a questa situazione e non limitarsi semplicemente alle promesse di un rinvio futuro. quindi che il Governo prenda questo impegno a mantenere inalterate quantomeno le risorse previste dalla legge n. 431.

Per riavviare tale mercato, si prevede una forma di incentivazione; ovviamente saremmo d'accordo con il Governo e il relatore a trattare gli importi, ma il principio ci sembra alquanto opportuno e interessante. Quindi chiediamo l'accantonamento

riguarda un tema molto semplice, che però è già oggetto di controversie giuridiche, e quando vi sono controversie giuridiche sostanzialmente si buttano soldi, in particolare Comuni e imprenditori.

Riteniamo che un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare la materia e a trovare una soluzione sia la via più opportuna.

quanto un decreto legislativo del 2006 aveva disposto in ordine all'asseverazione dei piani economico-finanziari per il *project* *financing* a favore degli enti locali.

come tempo addietro fu richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riguardo all'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 104. Il Garante, infatti, rilevava che il legislatore aveva ampliato lo spettro dei soggetti operanti sul mercato, prevedendo anche le società di revisione accanto agli istituti di credito. Sta di fatto che con una modifica, contenuta all'articolo 1, lettera *ee)*, del decreto legislativo n. 152 del 2008, è stata cancellata dal comma 9 dell'articolo 153 del precedente decreto legislativo n. 163 del 2006 l'attribuzione del potere di asseverazione dei piani economico-finanziari e della finanza di progetto alle società di revisione contabile operanti ai sensi della legge n. 1966 del 1939. Con l'approvazione di questo emendamento, che - si badi bene - non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, si ripristinerebbe la titolarità del potere di asseverazione anche in capo alle società di revisione contabile. Desidero aggiungere, d'intesa con il presidente Baldassarri e con il collega Fasano, che pure ha firmato l'emendamento in oggetto, che questa esclusione era del tutto immotivata e peraltro in completa dissonanza rispetto alla legislazione statale vigente e alle direttive europee, nonché alle citate indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza. Il presidente Baldassarri, il collega

oneri. Faccio un appello alla sensibilità di tutti presenti e del Governo in particolare. Il sottosegretario Casero conosce perfettamente questa vicenda e sa benissimo e sa benissimo che in precedenza c'era stata offerta una disponibilità ad andare incontro a questa necessità dell'Autorità,

a favore del bilancio dello Stato, rifiutiamo una sua accorata richiesta di consentirne una migliore organizzazione,

e chiedo a tutti la massima attenzione su questo aspetto.

ha bisogno di una risposta, perché i diritti non si misurano mai in base alla grandezza di un Comune o al numero di abitanti di una zona o alla consistenza della presenza parlamentare.

si è fatta una programmazione fino al 2033. Credo che anche questa comunità abbia diritto a una programmazione perché

bisogna dare delle risposte.

gli amici abruzzesi e il senatore Mascitelli ricorderanno - poiché essa è uno strumento di rinascita di aree povere. Non solo la zona franca urbana, abbiamo inventato la zona franca delle aree montane. Mi dite perché

*(PD)*. Signor Presidente, in una recente intervista, il Ministro della difesa ha affermato, con grande preoccupazione, che se non si modifica la situazione delle risorse per il comparto sarà impossibile reclutare i nuovi necessari volontari o mantenere in servizio quelli che stanno operando nei vari teatri di crisi. Ciò è la conseguenza del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha ridotto in maniera significativa le risorse per la professionalizzazione: cento nel 2009 e addirittura del 40 per cento nel 2010 e negli anni successivi. La riduzione del 2009, ancorché contenuta, ha già determinato una situazione di sofferenza; quella del 40 per cento sarebbe assolutamente penalizzante per le capacità operative dello strumento militare. Diventerebbe infatti impossibile mantenere il modello di difesa che il Parlamento ha approvato nel 2000, sulla base degli impegni delle Forze armate. impossibile rispettare i tempi per la riconfigurazione in senso professionale delle nostre Forze armate. Soprattutto, come ha denunciato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione del medesimo Ministero della difesa, si determinerebbe la perdita di potenziali e qualificate potenzialità. Ebbene, l'emendamento 2.561 intende evitare il suddetto taglio del 40 per cento e le sue gravi conseguenze, per dare alle Forze armate prospettive e possibilità adeguate ai compiti che esse sono chiamate ad assolvere. Chiedo pertanto alla maggioranza e a tutta l'Assemblea di sostenere tale emendamento, sottolineando che esso richiama esattamente quanto chiesto dalla Commissione difesa,

a limitare al solo 7 per cento la riduzione dei fondi destinati alla professionalizzazione delle Forze armate» per il 2010.

da vendite immobiliari. La proposta è il frutto di una considerazione supportata anche dall'afflusso che si sta verificando in virtù dell'istituzione dello scudo fiscale. Stanno rientrando le somme custodite nei conti correnti; quelle scaturenti da vendite immobiliari o da vendite di pacchetti azionari, invece, difficilmente rientreranno nei termini previsti dalla legge perché lo smobilizzo e la possibilità di consentire il rientro di tali somme sono più lenti per l'oggettiva difficoltà che si registra nella vendita di questo tipo di cespiti patrimoniali. Credo che l'emendamento produrrebbe un effetto di grande vantaggio per le casse dell'Erario sono convinto che non altererebbe l'andamento dell'attuale rientro perché questo, come dicevo, riguarda prevalentemente risorse custodite nei conti correnti, e quindi di facile smobilizzo e trasferimento

quella che è definita sommariamente «rottamazione del pubblico impiego». Un provvedimento di questo tipo consentirebbe un notevole risparmio per la pubblica amministrazione, ma soprattutto permetterebbe a molti Comuni e a molte amministrazioni pubbliche in genere (mi riferisco per esempio alla Sicilia, ma non solo) di collocare in questa forma di prepensionamento (che in realtà prepensionamento non è)

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'ordine del giorno G2.144 affronta una questione che personalmente reputo centrale e di assoluta importanza, ossia l'assetto proprietario della Banca d'Italia.

non può certo rimanere in capo a quegli stessi soggetti nei confronti dei quali si dovrebbe attivare la vigilanza. Infine, per assurdo, nel momento in cui i mercati subiscono un'azione forte e continua di penetrazione da parte dei fondi sovrani (in particolare cinesi e indiani), esiste

della Banca centrale europea. Credo, quindi, che vi siano tutte le condizioni per l'accoglimento di questo ordine del giorno, anche alla luce del dispositivo che lascia ampi spazi di manovra, in quanto recita: «impegna il Governo a dare attuazione, secondo le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, a quanto necessario e peraltro normativamente già stabilito, per riportare in mano pubblica la proprietà della Banca centrale italiana». Il riferimento legislativo è in particolare al comma 10 dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 2005, n. 262, che già prevede l'adozione di uno specifico regolamento per la ridefinizione dell'assetto proprietario e l'esclusione della parte privata.

in questi giorni dato il coro di proteste che si è levato dalle imprese e dai cittadini per chiedere al Governo di ritornare sulla propria Il nostro emendamento si propone di inserire, dopo l'articolo 2, un articolo 2-*bis* per istituire un fondo di circa 600 milioni (200 per ogni anno finanziario da qui al 2012) 2012) per cofinanziare progetti per lo sviluppo della banda larga nel nostro Paese: progetti per gli enti locali; progetti per i Comuni delle aree montane a bassa densità abitativa; progetti per lo sviluppo di reti *wireless* nelle aree urbane dedicate all'infomobilità e alla sicurezza dei cittadini, ai servizi per gli anziani e i disabili, allo sviluppo del turismo e ai beni culturali; progetti, infine, dedicati a favorire l'accesso a Internet delle piccole e medie imprese appartenenti ai principali distretti industriali. questo fondo, che noi avevamo pensato aggiuntivo agli 800 milioni del piano Romani, oggi rischia di essere l'unica possibile dotazione Per questa ragione noi chiediamo ai membri della maggioranza di ripensare alla questione e di votare per questo emendamento che può aiutare lo sblocco del progetto della banda larga nel nostro Paese. Noi vi prendiamo in parola: ci sono state tante dichiarazioni, a partire da quelle del ministro Scajola, favorevoli ad un ripensamento sulla decisione di bloccare i finanziamenti per la banda larga. Vi chiediamo di dimostrare nei fatti nei fatti che accogliete il senso delle proteste e che siete disponibili a cambiare atteggiamento. Per questo vi invitiamo a votare per il nostro emendamento. In caso contrario, il popolo della rete, le imprese gli italiani tutti avranno la conferma che questo Governo è ostile all'innovazione tecnologica, rema contro la competitività delle imprese e non ha idee e proposte serie per ammodernare il Paese e per far uscire più forte l'Italia dalla crisi economica. Per questo vi chiediamo di sostenere l'emendamento.

e beni alle stesse. Ormai i crediti delle piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono arrivati quasi a 40 miliardi di euro. Siamo in una situazione economica difficile e complicata,

cassa degli enti locali. Quindi, chiedo una riflessione profonda alla maggioranza su questo emendamento che potrebbe veramente dare un segnale vero e concreto alle imprese e al mondo economico, che lo aspetta da tempo.

la senatrice Serafini a proposito di politiche della famiglia. Vorrei sottolineare il fatto che noi siamo il Paese più vecchio in Europa, e nel mondo siamo superati solo dal Giappone; un Paese dove le attese di vita sono sempre più elevate: siamo a 73,2 anni di aspettativa di vita per gli uomini ed 83,2 anni I dati ci dicono addirittura che una bambina nata nel 2009 ha oltre 100 anni di aspettativa di vita, naturalmente alle condizioni attuali. È evidente a tutti che con l'aumento dei soggetti ultrasessantacinquenni, che costituiscono una percentuale sempre più elevata della nostra popolazione, sono in aumento anche le probabilità di diventare non autosufficienti. C'è già stato, per quello che riguarda il settore della sanità, un allarme circa l'esplosione della spesa. Eppure non c'è un programma di prevenzione della non autosufficienza, manca un'attenzione ad elaborare linee di intervento che riducano il più possibile il numero delle persone non autosufficienti. questa mancanza non è solo nella prevenzione, ma anche nel sostegno a quando ormai una persona è non autosufficiente. un finanziamento adeguato ad un fondo che, come veniva ricordato, nel 2010 sarà praticamente senza risorse. Questa mancanza di risorse fa sì che già attualmente le famiglie si debbono far della cura dei propri cari non autosufficienti: le Regioni e i Comuni non sono in grado oggi di rispondere ad una richiesta sempre più ampia di servizi, siano questi di carattere residenziale che di carattere domiciliare. Non a caso, nel nostro Paese, molta parte di questa assistenza è svolta da quelli che volgarmente vengono definiti badanti, anche persone che vengono dai Paesi comunitari ma con gravi situazioni economiche, che si accontentano di una

Accolgo molto favorevolmente quindi il fatto che nel Patto della salute sia stato per la prima volta inserito l'impegno ad attivare dei flussi informativi

per la salute, sottoscritto recentemente, vi è l'impegno del Governo a finanziare con 400 milioni di euro il Fondo per la non autosufficienza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ancora una volta richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su un tema specifico, di cui più volte ho parlato in quest'Aula: si tratta della tutela delle minoranze linguistiche, sia le diverse minoranze presenti sul territorio nazionale che quelle italiana e slovena in Croazia. Il Governo ha mostrato finora totale disinteresse verso questo tema, nonostante le diverse enunciazioni di principio. Il disinteresse del Governo si manifesta anche attraverso la finanziaria, visto che siamo al secondo anno in cui vengono drasticamente tagliati i fondi alle minoranze. Per quanto riguarda gli italiani in Istria, ci sono state a tale proposito le rassicurazioni del presidente Fini nel recente incontro con la delegazione del Parlamento croato, di cui faceva parte anche il deputato croato della comunità italiana Furio Radin. Rispetto agli sloveni del Friuli-Venezia Giulia vorrei ribadire che l'entità del finanziamento è prevista dalla legge di tutela n. 38 del 2001 e con questa finanziaria si viola anche tale legge. L'anno scorso si è operato nello stesso modo, salvo poi recuperare 1 milione di euro con la cosiddetta legge milleproroghe. Vorrei sentire un impegno concreto da parte del Governo, che possa dare le rassicurazioni necessarie alla comunità slovena per poter guardare con un certo ottimismo al proprio futuro. In questo momento ci sono segnali molto negativi: la grave crisi del teatro sloveno; la mancata applicazione di parti della legge n. 38; le preoccupazioni rispetto alla riforma della scuola. Se dovesse realizzarsi anche il taglio dei fondi, allora la situazione potrebbe diventare dirompente, ma soprattutto ciò significherebbe violare uno dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e dai trattati in ultima analisi, ciò non giova al clima di pacifica convivenza tra l'Italia e la Slovenia e tra l'Italia e la Croazia e non giova alla crescita comune di questa importante area dell'Unione europea, dove la presenza di diverse culture e lingue dovrebbe rappresentare un fattore di ricchezza e una sfida culturale. Mi auguro perciò che si possa arrivare a ripristinare i fondi della finanziaria 2008.

Signor Presidente, da molti anni si attende un intervento legislativo che possa disciplinare organicamente il settore delle case da gioco. Di fatto, la normativa vigente risulta contraddittoria ed incapace di disciplinare in maniera chiara ed omogenea la materia. Come è noto, in Italia, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale, che prevedono e sanzionano come ipotesi di reato l'esercizio di giuochi d'azzardo e l'apertura di case da gioco, esistono quattro casinò La stessa Corte costituzionale, rilevando i paradossi del sistema normativo, aveva a suo tempo sollecitato un intervento del legislatore e si è più volte pronunciata sulla questione, in particolare nella sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, nella quale ha affermato che «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità». Si impone quindi una legislazione organica di settore. Nelle ultime tre legislature numerosi parlamentari hanno presentato proposte di legge riguardanti il settore delle case da gioco. Nella XIV legislatura, tra Senato e Camera dei deputati, sono state presentate ben 54 proposte di legge; nella XV legislatura i disegni di legge sono stati 20,

del numero delle case da gioco e, nello specifico, sull'istituzione di case da gioco territoriali o stagionali allo scopo di risollevare l'economia turistica locale e, sull'introduzione di regole più uniformi, in un settore che, ad oggi, presenta numerose lacune. Durante la XIV legislatura, in particolare, nell'ambito del Comitato ristretto istituito durante i lavori della 10a Commissione permanente, è stato elaborato un testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco, testo che è stato recepito nella stesura dall'emendamento da me presentato unitamente ad altri colleghi. Più recentemente, come noto, a seguito dell'approvazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", divenuto legge il 23 giugno 2009, vi è stata una miniriforma dei giochi: all'articolo 12 del suddetto decreto vengono introdotti, infatti, nuovi giochi pubblici allo scopo

dalle agenzia di stampa, il ministro del turismo Michela Brambilla era in procinto di presentare al Consiglio dei ministri uno schema di decreto legge che intende rilanciare l'offerta turistica italiana. La bozza di testo, sempre in relazione alle suddette notizie, prevedeva, in particolare, l'apertura di case da gioco all'interno di strutture alberghiere almeno a cinque stelle. Tali ipotesi e proposte hanno lasciato dubbiose le organizzazioni del settore, che hanno evidenziato, oltretutto, la congiuntura particolarmente negativa, dovuta alla crisi economica e occupazionale, che le case da gioco stanno attraversando. L'emendamento 2.0.600 mira, quindi, a colmare la condizione di lacunosità che caratterizza la situazione normativa attuale per ciò che concerne l'istituzione delle case da gioco e l'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo. legislazione organica in materia si impone, oggi più che mai, anche per contrastare il fenomeno del gioco clandestino, unitamente ai fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, estorsione Appare chiaro che l'istituzione di nuove case da gioco controllate dallo Stato potrebbe porre un rimedio al ricorso, ormai sempre più preoccupante, al gioco di provenienza illecita. per evitare il proliferare di giochi d'azzardo mascherati sotto varie forme, come ad esempio le *slot machine*, i *videopoker*, eccetera, e per adeguare la legislazione alle linee di tendenza espresse dalla legislazione comunitaria. Infatti, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche eccezioni. Entrando nel merito del testo, l'emendamento 2.0.600 prevede che i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent possano proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo. Ulteriori Comuni, fino ad un massimo di otto, sono autorizzati all'esercizio dello stesso, sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale e a seguito dell'emanazione di un decreto da adottarsi entro 6 mesi da parte dei Ministeri competenti in materia. Tale decreto stabilirà le definizioni, le modalità, la durata, i divieti e la ripartizione dei proventi dei giochi ed, inoltre, nel prevedere l'individuazione dei Comuni autorizzandi, tenendo conto dei Comuni già già titolari di concessione e per ciò che riguarda i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale. È riservato, inoltre, alle società - questo è importante - che gestiscono le case da gioco attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco. Sarà poi compito del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, di emanare il regolamento di attuazione che si occuperà della previsione di specie, tipi e regolamentazione di giochi praticabili, delle disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e per controllare lo svolgimento del gioco stesso. In conclusione, tra tutte le proposte presentate fino ad oggi, quella contenuta in questo emendamento appare la più equilibrata e moderata, tenendo conto del fatto che, come detto precedentemente, il testo in esame ha recepito le linee generali contenute nel testo unificato sulla regolamentazione e istituzione delle case da gioco proposto dalla 10a Commissione durante la

l'emendamento 2.86 lanciamo ancora una volta una sfida e richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea, perché tocchiamo il classico tema, che da decenni si rincorre, relativo al ponte sullo Stretto. Il PdL ha voluto inviare un ulteriore segnale, molto di fumo e poco di sostanza, verso la realizzazione di questa infrastruttura. Noi diciamo invece all'Assemblea, al Parlamento e al Paese di fare attenzione perché il mondo, l'evoluzione dei traffici e dei commerci, lo spostamento delle persone, la viabilità richiedono un'altra collocazione del Paese a livello di priorità e anche di investimenti nel sistema delle infrastrutture.

ma chiede, in modo particolare, la possibilità d'investire sulle autostrade del mare e sulla infrastrutturazione dei corridoi del nostro Paese. A tal proposito, noi avanziamo qui una proposta di finanziamento per fare in modo che il nostro Paese sia ben organizzato per rispondere a quella evoluzione, a quella crescita, a quella diminuzione dei costi dei trasporti che solo attraverso un sistema intermodale,

per rispondere alle sfide della competitività mondiale e per beneficiare di un sistema moderno e avanzato di logistica dei trasporti. Ecco perché il nostro emendamento sposta le risorse, che ad agosto avete di nuovo buttato in questo calderone senza fondo, e le ricolloca negli assi, nelle strategie e nei corridoi, che sono appunto lì

dal ministro Tremonti nella finanziaria per il 2006. È uno strumento che ha dato risultati di grande e straordinaria importanza e rilevanza per il nostro Paese. In base agli ultimi dati disponibili, quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2008, circa 15 milioni di italiani (cioè più della metà di tutti i contribuenti) hanno destinato il 5 per mille ad organizzazioni *no profit*, per un importo che, sempre in base agli ultimi dati disponibili, è stato superiore ai 350 milioni milioni di euro, di cui sono state beneficiarie circa 30.000 associazioni di volontariato e utilità sociale. Gran parte di questo importo è andata al volontariato, ma una parte rilevante (63 milioni) è andata alla ricerca sanitaria e quasi 60 milioni alla ricerca scientifica. Ad oggi, la finanziaria per il 2010 non prevede il rinnovo di questo strumento. Tale fatto, senza contare i cronici ritardi nel pagamento del 5 per mille per gli anni scorsi, riveste una gravità

si riempie la bocca con la parola sussidiarietà: ebbene, queste associazioni, che si occupano di tante cose diverse (di assistenza sociale, di ambiente, di ricerca, di assistenza alle persone), svolgono funzioni che, ove se ne occupasse direttamente la pubblica amministrazione, costerebbero ai contribuenti molto di più. So che anche colleghi della maggioranza e del centrodestra - a cominciare dal senatore Gasparri, che si è occupato della questione - hanno chiesto la reintegrazione

del senatore Barbolini, possano essere accolti dal Governo e dalla maggioranza e che nei prossimi mesi, il più rapidamente possibile, lo strumento del 5 per mille esca da quell'incertezza che chiede poi, alla fine di ogni anno, in occasione di ogni finanziaria, di

trattandosi di un tema che non può prestarsi a logiche di schieramento - di fare uno sforzo straordinario, ottenendo dal Governo immediatamente il reintegro del 5 per mille per l'anno che sta per cominciare.

Vorrei raccomandare all'attenzione di quest'Aula che il provvedimento, già nei primi due anni di vita, quindi in una fase per così dire di sperimentazione e di avvio, ha permesso il risparmio di circa 2.800 gigawatt/ore di energia elettrica,

e che nella ristrutturazione trova il completamento migliore di quel sostegno, perché ovviamente si premia l'industria edilizia più innovativa, quella in grado di fare questi interventi che permettono il risparmio energetico.

poi il Governo ha dovuto recedere da quell'impostazione per la protesta delle associazioni ambientaliste, ma soprattutto delle imprese e dei cittadini, che in questo settore investivano, e quindi alla fine quel 55

riguarda gli ammortizzatori sociali cassa integrazione e disoccupazione. È inutile che parli del merito, perché è noto, sono anni che se ne discute ed è sempre sorprendente che, nonostante il consenso ampio (ci sono stati

ora più che mai un tema del genere va reso attuale, perché tutti i Paesi europei, anche quelli che hanno un sistema di ammortizzatori universali, li stanno rafforzando ed estendendo verso aree di lavoro deboli e di imprese deboli che sono dalla crisi messe a rischio. Sappiamo che la crisi, anche se quella produttiva sta finendo, per la parte occupazionale continua, quindi dovremo prendere in considerazione un intervento del genere. Non ha senso Non ha senso dire che non è il momento perché la crisi impedisce di fare degli interventi organici, perché si sa come un intervento di questo tipo può essere fatto (noi lo abbiamo discusso più volte senza costrutto) e si sa anche che può essere messo a regime progressivamente, il nostro è l'unico Paese d'Europa che non sta facendo niente in questo senso. Le casse in deroga hanno avuto un iniziale senso positivo:

E non lo dice solo la Banca d'Italia, che lo sostiene da tempo, ma anche inchieste di organi di stampa certo non sospetti proprio oggi sostengono che la gravità di molti casi scoperti è tale che c'è un milione di piccole imprese artigiane ed industriali che sono a rischio, che ci sono centinaia ci sono centinaia di migliaia di lavoratori (altro che posto fisso!) che stanno uscendo dalla protezione, magari sotto il titolo delle partite IVA:

a regime progressivamente. Per altri versi, possiamo pescare in diversi capitoli, e basterebbe sentire il collega Mario Baldassarri. Per questo motivo, insistiamo su tale emendamento.

Signor Presidente, desidero illustrare la proposta emendativa relativa agli incentivi per lo sviluppo del sistema dei Confidi nel Mezzogiorno. Si tratta dell'emendamento 2.0.2 che può realizzare una larghissima maggioranza di consensi, poiché, mentre ancora non si diradano le nubi relative all'annunciata Banca del Sud, attraverso un sostegno al sistema dei Confidi, dei consorzi di garanzia fidi e delle cooperative di garanzia, siamo in grado di rispondere in modo molto concreto ed efficace ad un problema gravissimo, che riguarda le piccole e medie imprese del nostro Mezzogiorno, e alla stretta creditizia che tutti conosciamo e denunciamo. In Commissione bilancio, durante le audizioni in vista della legge finanziaria, abbiamo potuto ascoltare il Presidente dell'ABI, il quale ci ha riferito incredibilmente di non riconoscersi in una grave stretta di credito per il Mezzogiorno. La realtà non è così:

come alle garanzie, in particolare per le piccole e medie imprese. Con questo emendamento - che potrebbe essere votato da tutta l'Aula del Senato, perché sono certa che tutti i senatori di maggioranza lo condividono - sosteniamo lo sviluppo dell'aggregazione del sistema dei Confidi. È un processo già in atto nel Mezzogiorno: finora i Confidi non si sono mai sviluppati,

fare in modo che almeno quest'anno serva alla cooperazione allo sviluppo e alla difesa della politica estera di questo Paese. Signor Presidente, i nostri emendamenti e un ordine del giorno che mi permetto di illustrare puntano soprattutto sulla promozione della famiglia e delle nascite.

Sappiamo tutti che il Governo era ed è obbligato ad aumentare gradualmente l'età pensionabile delle donne per portarla dai 60 ai

Questo significa che anche le donne in Italia dovranno arrivare ad un'età pensionabile più avanzata, cioè a 65 anni.

tra i più bassi d'Europa e del mondo - non riusciremo più a sostenere a lungo termine il sistema pensionistico, non riusciremo a sostenere a lungo termine il sistema sanitario non riusciremo a pagare le spese per le badanti e per le persone che diventano sempre più anziane. Questo perché una fascia sempre minore di giovani dovrà prendere

che i risparmi incamerati grazie all'innalzamento graduale dell'età pensionabile delle donne venissero nuovamente investiti sulla famiglia e sulle donne per promuovere la natalità

ad «equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna prevedendo una riduzione dell'età pensionabile per la donna per un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni». Ricordo a quest'Assemblea che già la legge attuale prevede per ogni figlio un'anticipazione dell'età pensionabile di quattro mesi. Mi sembra poco; mi sembra giusto aumentare questa misura, misura, non solo come aiuto sociale alle famiglie ma anche come aiuto alla sostenibilità del sistema pensionistico e sociale di questo Paese. l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 30 per cento; - la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali

Si chiede per esempio per i coltivatori agricoli diretti di poter aumentare liberamente il proprio contributo previdenziale per poter usufruire in età pensionistica di una pensione un po' più alta di quella prevista. Al momento infatti è stabilito un limite massimo del proprio contributo; non capisco perché si debba negare la possibilità di pagare di più per avere una pensione più alta.

Tra l'altro abbiamo provveduto a rendere volontaria e non più obbligatoria l'autocertificazione ai fini del DURC

Ebbene, mentre gli studenti italiani o coloro che studiano in Italia possono usufruire di agevolazioni fiscali non è possibile fare altrettanto per coloro che studiano all'estero. Mi sembra una palese disattenzione, oltre che un'ingiustizia.

un figlio è a carico solo se guadagna meno di 2.840,51 euro all'anno.

si è già impegnato, nei giorni scorsi, a provvedere gradualmente a un intervento in questo senso.

2.700, 2.500, 2.99, 2.103, 2.106,

2.246, 2.702, 2.703, 2.248,

di ore per l'assistenza; erogazioni degli ausili, soprattutto dei comunicatori, importantissimi per questi malati.

però ricordare che questi malati hanno veramente bisogno di assistenza e di fondi, perché le loro famiglie continuano a pagare cifre davvero esorbitanti (circa 1.500 euro al mese) per poter avere un minimo di assistenza che ancora lo Stato non riesce ad

guardando in faccia la realtà, ho ritenuto che fosse meglio uscire e ricominciare da capo una battaglia per il cambiamento della politica.

è un obbligo per tutti. Ecco perché nel Gruppo Misto oggi, nel rispetto assoluto dei colleghi, che ringrazio per la stima e l'amicizia che mi hanno dato, spero di poter lavorare nell'interesse della della nostra comunità e della mia comunità regionale, con un unico discrimine però: sono nato cattolico popolare e come tale

la mia dichiarazione di appartenenza. Oggi nel Gruppo Misto con questo recinto, domani chissà, con una forza politica nuova che mi possa permettere,

Signor Presidente, segnalo a tutti i senatori che nella casella di posta c'è una lettera dell'onorevole La Russa che ci informa di avere rilanciato nei giorni scorsi la proposta di invitare tutti i parlamentari e gli altri eletti a sottoporsi

mesi. Sappiamo da notizie stampa che anche il senatore Giovanardi, che poc'anzi era in Aula, ha lanciato la stessa iniziativa e bisognerebbe capire se si tratta della stessa. Da una parte, infatti, il senatore Giovanardi ha detto che l'iniziativa dall'altra invece il ministro La Russa, il cui Dicastero di tutt'altro si dovrebbe interessare, ha detto che chi aderirà all'iniziativa si impegna a consentire di rendere pubblico l'esito del test ed accetta che l'iniziativa abbia un comitato di garanti composto, niente di meno, da almeno tre giornalisti. Resta la pienezza della demagogia e del populismo di questa iniziativa. Invito i senatori che volessero sottoporsi a questo tipo di di test, che inizierà dal 12 novembre - se avessero mai assunto delle sostanze proibite negli ultimi sei mesi sono avvisati che vanno incontro da una parte al trattamento della tutela della *privacy*, dall'altra al pubblico ludibrio di associarsi alla richiesta di capire quale dei due parlamentari e rappresentanti del Governo è titolare di questa incredibile iniziativa, ma soprattutto di capire se a seguito della eventuale pubblicazione del risultato del test

Senatore Perduca, naturalmente il suo è un intervento legittimo, ma non può chiedere certo alla Presidenza di sciogliere il nodo dell'iniziativa. È un'informazione che lei ha voluto dare ai senatori e resterà al verbale la sua valutazione, dopodiché se vuole che sia sciolto il nodo,

sono intervenuti con spranghe ed altri strumenti non legittimi intimando agli operai che occupavano

di gravità inaudita sia per i lavoratori, sia per una situazione aziendale assai complessa che temo porterà a molti licenziamenti ed alla chiusura degli stabilimenti.

avrebbero la presunzione di avere una risposta da questo Governo. La prima riguarda la disponibilità - in una Regione dove non vi sono soldi per la sanità perché si sta pagando il debito sanitario - di un acceleratore lineare per la cura dei tumori, offerto da una società che paga il 75 chiede allo Stato o agli enti sottoposti di pagare il restante 25 per cento. Perché non si utilizza un'occasione simile per curare i tumori in una realtà dove tutto l'impianto sanitario, a causa del terremoto nell'aquilano, non esiste più?

finestra"). Senatore Lusi, posso dirle che la Presidenza sollecita costantemente il Governo per la risposta alle interrogazioni: lo stesso presidente Schifani ha scritto una lettera formale al Ministro per i rapporti con il Parlamento per richiamare l'attenzione sulla necessità che ci sia una risposta alle interrogazioni che hanno particolare urgenza e che sono state segnalate. Continueremo a farlo, magari anche in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Dopo mesi di silenzio, oggi vi è stato un incontro tra i sindacati e la FIAT sul tema della cassa integrazione, che non è andato a buon fine:

le gravi mancanze di anticipazione delle spettanze ai lavoratori e i problemi sulle garanzie per gli attuali organici in forza. Abbiamo la preoccupazione che si apra uno scenario molto pericoloso per i lavoratori di Pomigliano, Pomigliano, dopo mesi e mesi di cassa integrazione a singhiozzo, di mancanza di garanzie, di mancanza di una prospettiva sulla missione industriale di quell'impianto FIAT, di mancanza di incontri e di tavoli istituzionali. Presidente, glielo ripeto ancora una volta, abbiamo abbiamo presentato 4 o 5 interrogazioni sulla questione di Pomigliano. Lo diceva prima il collega Lusi ed è inutile che lo ripeta anch'io. È da un anno e mezzo che sono qui e non ho avuto alcuna risposta, né su questa né su altre questioni. Come Gruppo del Partito Democratico presenteremo un'interrogazione non solo su Pomigliano, ma anche sulle altre aziende in crisi in settori strategici della regione Campania, quali la cantieristica e il tessile, oltre all'*automotive*. La presenteremo e porteremo qui ancora una volta la sofferenza e la difficoltà dei lavoratori.

per manifestare (per quanto possa essere importante, ma tale è per la mia coscienza) la mia profonda indignazione per gli epiteti

Cucchi, apostrofandolo con le espressioni "drogato", "sieropositivo" e "anoressico". Tutto questo credo sia inquietante. Tutto questo trovo rappresenti la cifra di un imbarbarimento che non può essere consentito neppure al più distante dalle normali consuetudini con il diritto e con la *pietas* e che tantomeno può essere accettato quando viene espresso da un uomo di Governo. Nel veder girovagare questa sera il sottosegretario Giovanardi ho avuto la speranza che fosse venuto qui per proporre uno strappo procedurale, magari perché colto da un irrefrenabile bisogno di chiedere perdono. Invece questo non è accaduto. Allora io vorrei, signor Presidente, che senza esercitare atteggiamenti, o di paternalismo o di censura, nei confronti di quest'uomo, si trovasse almeno il modo per rivolgersi a Stefano Cucchi manifestandogli rispetto, riconoscendogli, se era drogato, il diritto delle proprie scelte, e se era anoressico o sieropositivo, il diritto della propria malattia; e nell'occasione, Presidente, chiedere al Sottosegretario se alla stessa stregua di Tito, crocifisso insieme a Dimaco a fianco a Gesù, non sia il caso di cimentarsi per cercare l'amore superando la pietà che non cede al rancore. Avere un Sottosegretario di questo lignaggio è un problema, non soltanto per le istituzioni, ma anche per le coscienze e se questo signore non dovesse decidere di andar via per ciò che ha fatto, sarebbe bene comunque che, anche a mezzo posta, facesse pervenire alla famiglia di Stefano Cucchi e quindi agli italiani che di questa notizia hanno avuto coscienza le proprie scuse più profonde affinché queste cose non si verifichino mai più.

che lei sottolineava.

Signor Presidente, intervengo per sollecitare ancora una volta il Governo, a mezzo della Presidenza del Senato, affinché fornisca una risposta alle ormai tante interrogazioni che da questa primavera in poi sono state presentate dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico circa le condizioni di prechiusura delle imprese che operano in Italia nel settore dei metalli non ferrosi. Colgo l'occasione di questa sera, perché stamattina la città di Cagliari è stata occupata dagli operai dell'Alcoa, che producono l'alluminio nel Veneto e in Sardegna per tutta l'Italia.

negli aerei. Ciò è dovuto al fatto che non arriva una risposta del Governo sul tema di come trattare la questione del caro energia per le produzioni energivore di questi metalli non ferrosi. è una questione come tante altre. No! Oggi la nave che arrivava da Civitavecchia non ha potuto attraccare a Cagliari perché occupata dagli operai dell'Alcoa, disperati per la perdita del posto di lavoro, che ne hanno impedito l'attracco. Analoghe Analoghe situazioni si vivono a Porto Marghera, nel Veneto, come sa bene il collega Stradiotto che ha sottoscritto con me l'ultima delle interrogazioni. Il Governo deve venire e rispondere di questo. È una questione che sta diventando non solo di competenza del ministro di competenza del ministro Scajola ma anche del ministro Maroni, se non si interviene. Noi non siamo in grado di reggere il colpo di una crisi che vede *d'emblée* sparire un settore produttivo. A Bruxelles, in queste ore, il Governo dovrebbe essere impegnato ai massimi livelli e non lo sta facendo - nel fronteggiare *lobby* di altri Paesi ed interessi macroscopici che intervengono nella determinazione anche di questi aspetti delle politiche industriali. Ci sembra invece che esso sia totalmente distratto

circa il compito e l'esercizio della funzione di Governo da parte di chi ha ricevuto la fiducia del Parlamento. Non è più possibile tollerare il fatto immersi e sommersi dai decreti-legge, chiamati alla frusta e alla stanga a fare i legislatori a *jukebox*, mentre sulle questioni di indirizzo

principali per fare in modo che il Parlamento si occupi di simili temi, che stanno evidenziando ovunque in Italia le preoccupazioni di chi lavora e le tensioni della popolazione.